e sull'interessamento del COPASIR per la vicenda della signora Shalabayeva. Siccome non abbiamo notizie di tali accordi o protocolli riservati, vorremmo sapere se fosse possibile condividere queste informazioni con il resto dei colleghi,

Signor Presidente, colleghi senatori, se dovessi risultare sgradevole, sappiate che non è mia intenzione. Vorrei ribaltare un famoso *incipit* dicendo che tutto, fuorché la cortesia, mi porta contro questa proposta di legge. Il mio dissenso comincia dal titolo, si alimenta dal testo e diventa totale sull'idea stessa di toccare la Costituzione. Per rispetto del mio partito non voterò contro, ma, nel rispetto dell'articolo 67, non posso votare a favore. D'altronde, c'è già troppo unanimismo: si propagano luoghi comuni che sembrano veri solo perché ripetuti con sicumera dall'inizio, trent'anni fa. Il mondo è cambiato, ma l'agenda è rimasta sempre la stessa. L'entusiasmo iniziale delle bicamerali si è tramutato in una vera ossessione a modificare le istituzioni, una malattia solo italiana, che non trova paragoni in nessun altro Paese occidentale. È difficile credere che la nostra Carta costituzionale sia tanto più difettosa delle altre da meritare questo accanimento terapeutico. È più probabile che il malanno dipenda dagli improbabili costituenti. Siamo chiamati a dichiarare che la revisione della Costituzione è oggi una suprema esigenza nazionale. Mi chiedo perché, per che cosa e in nome di chi. La domanda sul perché riguarda la decisione. Si ricorre all'ingegneria istituzionale per obbligare il politico a fare ciò che non gli riesce spontaneamente, ma questo cadornismo applicato all'ordinamento è sempre fallito: il bipolarismo doveva eliminare la corruzione; il federalismo doveva promuovere lo sviluppo locale; il maggioritario doveva garantire la stabilità. Per dirla con don Abbondio, chi non ha la volontà politica, non se la può dare con gli artifici istituzionali. Eppure questa illusione è dura a morire. Ha sostenuto strategie politiche, ha animato i *talk show*, ha creato perfino il nuovo ordine professionale degli ingegneri istituzionali, costituito dai parlamentari esperti del tema - ai quali va comunque la mia stima personale - dai giuristi, che ne hanno fatto una carriera accademica, e dagli editorialisti, che ne hanno fatto una fortuna mediatica. L'ordine degli ingegneri si pone solo domande tecniche, ma il dato saliente del trentennio è la crisi dei partiti. La causa politica dell'ingovernabilità è stata trasferita in capo alle istituzioni. Se non si decide, non è colpa mia, ma dello Stato che non funziona: questo è il motto del politico, a tutti i livelli. Lo sviamento, però, non è stato innocuo: è servito come alibi alla politica per non affrontare i suoi problemi, che si sono di molto aggravati. Le istituzioni sono state stravolte per finalità di parte, invece di essere curate nella loro essenza. La promessa era di riformare lo Stato per migliorare i partiti, ma sono peggiorati entrambi; mai erano giunti tanto in basso nella stima dei cittadini. È tempo di fare sobriamente la nostra parte, lasciando in pace le istituzioni. L'unica riforma veramente necessaria è cambiare i nostri partiti per renderli adeguati al compito di governo del Paese. La domanda sul che cosa si è ridotta ad un mantra: il mondo cambia e bisogna decidere in fretta. Ma in quest'Aula sappiamo bene che le leggi più brutte sono proprio quelle più frettolose: il "porcellum" fu approvato in poche settimane; le leggi *ad personam* di gran carriera; diversi decreti di Monti, approvati con lo squillar di trombe, sono oggi smontati dal Governo Letta. Il decisionismo senza idee ha prodotto un'alluvione normativa che soffoca l'economia e la vita quotidiana dei cittadini. Ce la prendiamo con la burocrazia come se fosse un destino cinico e baro, ma invece essa dipende dalle troppe leggi che approviamo qui. Aveva ragione Luigi Einaudi a fare l'elogio della lentezza parlamentare come antidoto all'ipertrofia normativa. Non è la velocità ma la qualità che manca al procedimento legislativo. La causa è nello strapotere dei Governi che da tanti anni propongono solo leggi *omnibus*, con centinaia di commi disorganici, improvvisati, spesso modificati prima di essere applicati. Questa peste normativa distrugge l'amministrazione dello Stato, crea i contenziosi, le interpretazioni fantasiose e la paralisi attuativa. Bisognerebbe restituire al Parlamento la piena sovranità legislativa, ma questa autoriforma dovremmo farla noi, cari colleghi, senza delegarla all'ordine professionale degli ingegneri istituzionali, dovremmo attuarla con l'orgoglio di parlamentari: poche leggi l'anno, in forma di codici unitari, delegando funzioni al Governo e aumentando i poteri di controllo. Stabilire che non si legiferi senza prima valutare i risultati delle leggi precedenti. Dare alle Commissioni parlamentari poteri di inchiesta: un dirigente di Finmeccanica deve temere un'audizione come un *manager* americano quando va in Senato. Alla terza domanda (in nome di chi?) si risponde: nell'interesse nazionale. Eppure, ogni volta che abbiamo modificato la Costituzione ce ne siamo dovuti pentire: il Titolo V ha creato conflitti permanenti tra Stato e Regioni; dopo lo *ius sanguinis* del voto all'estero oggi si passa ad invocare lo *ius soli* per i figli degli immigrati; prima si blocca il pareggio di bilancio e poi si esulta per la deroga concessa dall'Europa. D'altro canto, basta leggere il testo per notare la differenza. La bella lingua italiana, con le parole semplici e intense dei Padri costituenti, viene improvvisamente interrotta da un lessico nevrotico e tecnicistico, scandito dai rinvii a commi, come un regolamento di condominio. Sono queste le parti aggiunte da noi. Fortunatamente i cittadini hanno evitato i guai peggiori bocciando la legge costituzionale ideata dagli stessi autori del "porcellum". L'unico baluardo è venuto dai presidenti di garanzia come Scalfaro, Ciampi e Napolitano. Mi sconcerta la leggerezza con la quale si ritiene possibile demolire questo ultimo bastione. In Italia la personalizzazione si è sempre presentata come patologia e non come responsabilità delle *leadership*. Non scherziamo col fuoco: il presidenzialismo non sarebbe un emendamento, ma un'altra Costituzione. Dovremmo avere un senso del limite. I nostri partiti rappresentano oggi a malapena la metà del corpo elettorale, l'altra metà ha manifestato in tutti i modi il disagio e la sfiducia. Noi non siamo quindi in grado, in questo momento, di rappresentare l'unità nazionale. Non è saggio usare la revisione costituzionale per santificare un Governo privo del mandato elettorale. Questo è il *vulnus* che segna la modifica Il procedimento lega la sorte del Governo ai tempi e ai modi della revisione costituzionale. Porre un vincolo di maggioranza come inizio e come fine nella della riforma è una forzatura politico-costituzionale senza precedenti in Italia e in Europa. I Governi passano, le Costituzioni rimangono, non dimentichiamolo. Dovremmo prendere atto che la nostra generazione non è capace di fare queste riforme, che possa farlo oggi al minimo storico del consenso elettorale è un ardimento senza responsabilità, è una dismisura contro lo spirito costituzionale. Lasciamo alle generazioni successive il compito di rielaborare l'eredità ricevuta dai Padri costituenti. Non tutte le generazioni hanno l'autorevolezza per cambiare la Costituzione. Dovremmo prenderne atto con umiltà, con l'umiltà di cui parla Papa Francesco, che dovrebbe sempre accompagnare l'esercizio del potere. La nostra umiltà è il migliore contributo che possiamo portare oggi alla Carta costituzionale. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge costituzionale che ci accingiamo ad esaminare e sul quale siamo chiamati a deliberare ci è stato, com'è noto, presentato dal Governo all'esito della composizione della crisi seguita alle ultime elezioni politiche. Non devo ricordare, se non a me stesso, le circostanze davvero inconsuete che hanno portato alla situazione presente: la difficile lettura del risultato uscito dalle urne, il per lui non felice passaggio del preincarico di formare l'Esecutivo ricevuto dall'allora segretario del Partito Democratico, la scelta del Quirinale di far decantare il clima politico investendo due comitati di esperti del compito di effettuare un rigoroso inventario delle urgenze del Paese, nel contesto della grave crisi economica che purtroppo ancora ci attanaglia e di fronte alle attese dei mercati, della comunità internazionale e delle istituzioni dell'Unione europea. Né lo stesso contesto geopolitico del Mediterraneo, cui apparteniamo per naturale collocazione, si è da quei giorni schiarito, preoccupandoci oggi per le notizie che ci giungono dal vicino Egitto. Quando in seduta comune con gli onorevoli deputati abbiamo - ed anche questo è stato un *unicum* della storia repubblicana - rieletto il presidente Napolitano quale Capo dello Stato, proprio da noi chiamato a succedere a se stesso a costo di vincerne la ritrosia chiaramente manifestataci, siamo stati tutti testimoni della severità del messaggio con il quale, nell'Aula di Montecitorio, ha accolto la rinnovata investitura. Egli ci ha, con la sua autorevolezza, esortato - e lo abbiamo applaudito anche per questo motivo - a non frapporre ulteriori ostacoli al necessario processo di riforme costituzionali ed elettorali, facendo prevalere il bene comune e la visione, finalmente resa concreta, di una rinnovata democrazia sulle piccole e reciproche polemiche quotidiane. Il presidente del Consiglio Letta ne ha puntualmente condiviso e assecondato i moniti, ribadendo per parte sua l'urgenza delle decisioni da assumere. Decisioni di indirizzo politico sì, ma anche e innanzitutto di quadro costituzionale ed istituzionale, entro il quale il primo dovrà esprimersi ed essere sorretto da una maggioranza che nessuno,

nel sostenere il disegno di legge costituzionale che oggi è al nostro esame, di corrispondere ad un mandato che è per me vincolante, nel senso di sollecitare le mie corde più profonde di parlamentare, ma prima ancora di cittadino e di padre, perché è ai nostri concittadini, a quelli che hanno votato ciascuno di noi, ma anche agli altri, e ai nostri figli, che dobbiamo mostrare di avere reale consapevolezza della gravità del momento che viviamo. Noi, e prima di noi il Comitato dei quaranta, chiamato ad esercitare in sede referente congiunta il compito di istruire le proposte di revisione costituzionale sulla forma di Governo e la struttura del bicameralismo sinora perfetto, o *a latere* gli esperti chiamati a fornire consulenza al Governo e al Ministro per le riforme istituzionali, non siamo destinati ad esercitare domani un potere costituente. Il compromesso costituzionale del 1948, sul quale seppero convergere i Padri della Repubblica, non sarà toccato nell'ordito mirabile dei valori e dei principi della sua prima e ancora vivissima parte. Questo mi piace ricordarlo, ponendo l'accento su questo aspetto, ad alcuni oratori, in particolare il senatore Giarrusso, che stamani è intervenuto parlando parlando quasi di uno sconvolgimento dei valori della Carta costituzionale. Senatore Giarrusso, non è così. Non è infatti ignoto che da sempre la dottrina costituzionale ha rivelato uno iato, un distacco, tra le innovatività e la capacità di implementazione inscritte in quei medesimi principi (di cui alla parte I della Costituzione) e la timidezza dell'impianto della parte II, scritto in tempi nei quali si facevano sentire differenze reciproche tra contrapposte forze politiche e il clima della guerra fredda. Siamo dunque chiamati non a stravolgere la Carta costituzionale, ma proprio ad adeguarne la parte propriamente organizzativa, affinché quegli ideali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà possano irrobustirsi e vivere anche nella nostra difficile epoca e nel futuro che impone, in presenza di una competizione globale, decisioni sì democratiche e il più possibile condivise, ma innanzitutto rapide. Non si indebolisce la Costituzione, per avanzare qui una decisiva osservazione tecnica, ma si articola diversamente la sua rigidità, con procedure eccezionali rispetto a quella attuale, di cui all'articolo 138 della Costituzione, agendo sui tempi del procedimento di revisione ma senza impedire in assoluto spazi spazi per emendamenti e ripensamenti e, men che mai, l'esercizio di eventuali questioni pregiudiziali. Apprezzabile risulta essere poi il criterio per la composizione del Comitato. Infatti non è prevista come usuale la composizione in maniera proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari. Provvidamente è previsto che si tenga conto anche dei voti conseguiti nell'ultima tornata elettorale dalle liste riconducibili ai singoli Gruppi. Gruppi. In tal modo è mitigata l'alterazione della rappresentanza politico-parlamentare determinata dall'attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla vigente legislazione elettorale (specie alla Camera) rispetto agli effettivi orientamenti espressi dal corpo elettorale. In effetti, il disegno di legge, per quanto possibile, si allinea alle acquisizioni più avanzate della riflessione costituzionalistica. In questo solco si allinea anche la previsione di chiamare il popolo sovrano a suggellare comunque, anche oltre i limiti previsti dall'attuale articolo 138, il risultato auspicato del procedimento di revisione costituzionale, ovvero eventualmente a respingerlo. Né va sottovalutata l'ampia e innovativa consultazione telematica che, a far data da ieri, impegnerà la partecipazione di chiunque voglia fornire il proprio contributo sui temi della riforma costituzionale e di quella elettorale, coerente con il disegno sortito dallo sforzo comune di esperti del suddetto Comitato e delle Assemblee che restano ciascuna autonoma e libera nelle proprie determinazioni. Se non siamo chiamati a disegnare la Costituzione, ancor meno ci è conferito il compito di scrivere la migliore astrattamente possibile. Dobbiamo però consentire che dopo almeno un trentennio di defatiganti discussioni, di intensi ma inconcludenti dibattiti riformatori (cui anche - ahimè - l'accademia ha dato il proprio apporto), dopo il nulla di fatto in comitati e commissioni bicamerali, il cui confronto è finito del pari in un vicolo cieco, si compia finalmente un percorso che, del resto, era apparso già maturo e per ampi tratti largamente condiviso nella scorsa legislatura, e tale è stato riconfermato con l'approvazione da parte delle Camere, lo scorso 29 maggio 2013, delle mozioni sulle riforme costituzionali. Con questo spirito, allora, dichiaro il voto favorevole in quest'Assemblea al disegno di legge costituzionale oggi in discussione, sereno: sereno di fronte alla mia coscienza personale e a quella della Nazione, concetto, quello di Nazione, che, come è a voi tutti noto, comprende anche chi è vissuto prima di noi

(opportunamente aggiornato nella forma, perché le eredità non devono essere rendite sterili, ma devono essere investite e fatte fruttificare), fruttificare), avrò contribuito a raccogliere e ad arricchire la speranza di libertà, giustizia e democrazia che i Padri costituenti consegnarono, perché durasse, al Paese, all'atto di riscattarlo dalla dittatura e di risollevarlo dalle immani distruzioni belliche.

senatori, oggi si dà avvio, mediante questo provvedimento, all'accensione della macchina delle riforme sostanziali, quelle costituzionali, quelle che per anni hanno suscitato poderose levate di scudi da parte delle caste e degli ordini precostituiti che da questo sistema di norme hanno tratto una linfa troppo esosa per le nostre tasche, e che non possiamo più permetterci sia in termini politici, ovvero di reale compiutezza della democrazia,

Da ogni parte, ogni settore imprenditoriale e produttivo, ogni categoria professionale italiana, tutto l'asse essenziale dell'economia del Belpaese, con le sole eccezioni - dicevamo - di qualche corporazione ormai lontana dalle esigenze e dalla storia di questa comunità nazionale, invoca un forte cambiamento nella struttura portante di questo insieme di norme che regola il vivere civile italiano. Non bisogna essere dei fini giuristi per capire che le modalità con le quali si sta mettendo in atto il meccanismo di innovazione giuridica costituzionale appaiono di gran lunga anomale e irrituali. L'importanza della materia di cui si discute, la delicatezza e la complessità degli argomenti trattati dal disegno di legge in esame ci inducono ad assumere una posizione di osservazione collaborativa, quindi ci spingono ad un'apertura di credito non incondizionata, ma di tipo fiduciario "a termine", nei confronti di chi ha ipotizzato questo tipo di soluzione legislativa. Non ha certo entusiasmato sapere che ci sarà un Comitato bicamerale di tanti rappresentanti, che dovranno confrontarsi su ogni cavillosa interpretazione del disposto costituzionale, spesso addentrandosi in sterili elucubrazioni dottrinarie ed accademiche, ma se questa è la strada che anche il nostro Presidente della Repubblica intravede per giungere al di là del tunnel, ebbene, non ci resta che far da guardiani del faro agli innovatori della nostra Costituzione. Per questa serie di motivi credo che non bisogna fasciarsi le testa se si vuole procedere, in deroga all'articolo 138 della Costituzione, ad intraprendere una via che agevoli il processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento e col fine di operare una innovazione sostanziale che vada nell'interesse del Paese e dei cittadini, per troppo tempo ostaggio di vecchie gabbie di leggi fuori dal tempo. È davvero apprezzabile la prontezza e il senso del rispetto che il Governo ha tenuto nei confronti dei cittadini comuni dopo che la Consulta ha bocciato la proposta di svuotamento e riordino delle Province contenuta nel cosiddetto decreto salva Italia. L'approvazione il giorno dopo di un disegno di legge costituzionale che avesse lo stesso oggetto è una risposta incisiva di questo Esecutivo ed è un chiaro esempio di come in Italia ci siano alcuni involucri legislativi che possono tentare di fermare un improcrastinabile processo di necessario cambiamento dello Stato; ma quando c'è una precisa volontà di far qualcosa che tutti gli italiani si aspettano, allora non c'è organo conservativo che tenga, soprattutto quando non solo la voglia di cambiamento è così diffusa nel senso comune dei cittadini, ma anche le esigenze culturali, il quadro sovranazionale e le contingenze socio economiche ce lo impongono. Di conseguenza, elaborato nella congiuntura cosiddetta delle larghe intese, questo provvedimento rappresenta una delle ultime opportunità che ha questa maggioranza di legittimarsi agli occhi della gente.

a differenza delle altre grandi democrazie dell'Occidente, che da tempo hanno messo in sicurezza le loro istituzioni costituzionali, il nostro Paese si è trovato, in un momento di profonda crisi economica e sociale, privo di strumenti adeguati alla portata delle decisioni da assumere. L'Italia, quindi, paga il prezzo del ritardo della modernizzazione dell'assetto istituzionale dello Stato e questo è insostenibile nella situazione in cui ci troviamo, non potendo noi permetterci di avere istituzioni inadeguate all'assunzione di decisioni, soprattutto tempestive. Questa è la sfida che abbiamo di fronte il disegno di legge costituzionale che discutiamo oggi deve quindi muoversi in questo senso, affinché aiuti ad individuare l'assetto istituzionale che meglio possa aiutare il Paese ad uscire dalla crisi politica e decisionale in cui si trova, secondo forme, tempi e modalità certi. Non si può continuare a tergiversare, a posticipare, a seguire particolarismi e localismi, a rimandare il problema a chi verrà dopo di noi: è troppo tempo che si fa cosi e non è giusto. Non dimentichiamoci che i nostri Padri costituenti hanno impiegato in tutto (comprese le proroghe) lo stesso tempo, cioè circa diciotto mesi, per scrivere ed approvare definitivamente la nostra Carta costituzionale. La situazione attuale ci chiede delle decisioni forti, che rispondano adeguatamente al bisogno profondo di riforme che il nostro Paese chiede. L'idea di fondo che hanno molti nostri concittadini, soprattutto le nuove generazioni, gli universitari e i giovani lavoratori, è che l'Italia sia ormai un Paese vecchio, fermo, immobile nella propria struttura, incapace per questo di andare avanti, di guardare al futuro, di cogliere ed offrire opportunità. È un Paese che toglie il respiro a chi ha voglia di fare, allontana la fiducia e, troppo spesso, la stessa volontà di fare a chi, come i nostri giovani, dovrebbe invece essere in prima linea nel costruire il nostro Paese. Per questo motivo molti di quelli che hanno e sentono il forte desiderio di fare si ritrovano a dover andare all'estero, oppure rinunciano, scontrandosi con una condizione politica, sociale ed economica e con un immobilismo che spezza i loro desideri e le loro ambizioni. La frustrazione ed il lamento diventano il sottofondo di ogni nostra azione. Perché siamo diventati un Paese incapace di riformarsi? Perché dobbiamo costringere chi ha voglia di costruire a dover guardare altrove, invece di partecipare attivamente al bene del Paese, al bene di tutti? Questo preoccupante immobilismo è figlio, purtroppo, anche di quello della politica, del nostro immobilismo. Se non ci affrettiamo a dare una risposta alle necessità di riforme di cui l'Italia ha disperatamente bisogno, avremo perduto l'ennesima occasione di costruire e di servire il bene del nostro Paese di dare almeno un principio di speranza, una spinta, a chi queste riforme ci chiede per il proprio futuro. Che immagine abbiamo potuto dare ai nostri giovani, che rappresentano il futuro, durante l'ultima elezione del Presidente della Repubblica? È fondamentale che ci poniamo domande come questa. Come si può sperare che tutti partecipino attivamente al progresso dell'Italia, se poi noi siamo i primi ad accontentarci, a non cambiare, stroncando cosi sul nascere tutta la buona volontà di molti che vorrebbero poter, con il loro fondamentale contributo, cambiare in meglio il Paese? Diventa quindi fondamentale la prontezza delle nostre proposte e del nostro lavoro e in questa direzione va il disegno di legge che oggi discutiamo e voteremo, il quale delinea, positivamente, scadenze e tempi certi per la discussione, il voto e l'approvazione, dato che non possiamo permetterci il lusso di tergiversare. Rispettare quindi i tempi definiti nella proposta è prioritario perché il nostro lavoro dia frutto e risposte concrete. il disegno di legge costituzionale che andremo a votare permetterà di creare le basi ed il terreno fertile per quelle riforme che assicurino la stabilità e la governabilità dell'Italia in questo momento di profonda crisi, sperando che siano solo l'inizio di un profondo rinnovamento, non solo istituzionale, ma anche economico, sociale e culturale del Paese, affinché esso

quello che oggi è all'esame dell'Aula è un disegno di legge inerente alle riforme non solo costituzionali, ma istituzionali. Un complesso di riforme che riguarda un più ampio arco di istituti: dalla legge elettorale all'assetto del bicameralismo, dall'equilibrio e controllo tra poteri e organi dello Stato alla riforma e al rinnovamento dei Regolamenti parlamentari. Siamo nella fase in cui si delinea il percorso per arrivare alle riforme costituzionali e il pensiero corre, necessariamente, alle parole pronunciate dal presidente Giorgio Napolitano nel suo discorso alle Camere in occasione del suo insediamento. La rielezione del Presidente della Repubblica non trova precedenti nella storia, ma è stata necessaria per superare il difficile stato di *impasse* creato dal risultato elettorale sì, ma anche da un atteggiamento definito come irresponsabile e di chiusura da parte di fazioni che non hanno inteso creare le premesse per la formazione di un Governo. Parole severe, le sue, chiare e di richiamo alla responsabilità di tutti noi parlamentari. Non possiamo pensare a un rinnovamento della classe politica, dei partiti, se non cambia - prima di ogni altra cosa - l'approccio alle gravi difficoltà in cui versa il Paese. Non si possono anteporre il perseguimento di tatticismi, la ricerca di convenienze, l'attuazione di strumentalismi, alla volontà di ricercare, con il buonsenso, la strada che ci può condurre alla governabilità, alla stabilità economica, a una prospettiva di crescita. Vogliamo un cambio generazionale? Il Parlamento è stato rinnovato in una sua parte consistente: si è abbassata l'età media, è più numerosa la presenza femminile, ma adesso dobbiamo anche dare la dimostrazione che il cambio di passo lo si vuole realmente! Un passaggio essenziale riguarda la legge elettorale. Come è noto la legge n. 270 del 2005, il cosiddetto "porcellum", ha ricevuto da più parti profonde critiche per gli effetti che ha prodotto e continua a produrre nel sistema politico italiano. Dalle urne, il 24 e il 25 febbraio scorsi, non è uscito un risultato chiaro, una maggioranza univoca che consentisse ad una forza politica di governare. Questo perché la legge elettorale del 2005 ha prodotto effetti diversi nei due rami del Parlamento: un premio a base nazionale alla Camera dei deputati e un premio a base regionale al Senato hanno determinato il paradosso di produrre due maggioranze diverse. Il risultato - lo abbiamo visto - è stata la grave situazione di stallo politico-istituzionale che ha attraversato il Paese prima della formazione dell'attuale Governo. Un immobilismo grave e pericoloso che assolutamente non dovevamo e non potremo più permetterci nella situazione di grave crisi economica in cui versa il Paese. Il Presidente della Repubblica, anche su questo argomento, ha richiamato la politica alla responsabilità definendo come «imperdonabile» il fatto di non aver riformato la legge elettorale del 2005. Tutti noi ci auguriamo di non dover più ricevere un così grave appello a muovere dei passi significativi e celeri per il superamento del cosiddetto "porcellum". Per questo credo che il tema della riforma elettorale debba essere una priorità, non solo per il Partito Democratico, ma anche per le altre forze politiche. Dobbiamo interrogarci su quali sono stati i *vulnus*, i punti deboli dell'attuale legge, cosa implicherebbe una sua correzione minimale - come da più parti si è vociferato - e cosa comporterebbe invece un ritorno d'emergenza al "Mattarellum", che pure tanti hanno invocato. Il Partito Democratico ha fatto la propria parte nel tentativo di superare la legge del 2005 attraverso le primarie per la scelta dei candidati. Ora dobbiamo scegliere davvero, e dobbiamo farlo in Parlamento senza ulteriori dilazioni temporali. La legge elettorale non deve essere un argomento tabù, come pure il bicameralismo perfetto. Ho condiviso, signor Ministro, le sue considerazioni in seno alla 1a Commissione a proposito degli effetti anche economici delle riforme costituzionali di cui ci attende l'elaborazione. In un'Italia in cui c'è urgenza di riforme, di risposte immediate alla crisi finanziaria, alla recessione, al malessere sociale, occorre prima di tutto un'analisi dell'attuale sistema, che, pur mettendo al centro il Parlamento, deve sistematicamente ricorrere alla decretazione d'urgenza per conseguire in tempi brevi il risultato atteso. Sono perfettamente consapevole che siamo ancora in una fase anteriore a tali scelte, ma non dobbiamo temere, sin d'ora, di avviare un dialogo costruttivo tra le forze politiche in merito al bicameralismo, ai Regolamenti parlamentari, alla legge elettorale. Negli ultimi mesi il tema delle riforme costituzionali è stato all'attenzione di tutti e, per questo, credo che dovrà interessare tutti il focalizzarsi anche sull'ipotesi di riforma del Senato come Camera delle autonomie. Un Senato eletto su base regionale, come già l'articolo 57 era stato pensato dai Padri costituenti, da ripensare nella più ampia cornice degli enti territoriali fissati dall'articolo 114. Un Governo della Repubblica e non dello Stato; un Governo e un Parlamento di concerto, che rappresenti e dia voce a tutte le realtà territoriali del Paese. Ritengo quindi che il momento di riforma che ci si prospetta davanti possa essere un buon momento di «rinnovamento nella tradizione», non di rivoluzione ma di manutenzione costituzionale più che di riscrittura della Carta. Interventi precisi, mirati, che assicurino rapidità, efficacia ed efficienza all'azione parlamentare. Le riforme devono servire a migliorare l'assetto istituzionale, innanzitutto per superare le prassi degenerative degli ultimi anni: dai decreti-legge *omnibus* alla continua apposizione della questione di fiducia da parte del Governo (magari su testi blindati con maxiemendamenti), all'abuso di decreti-legge anche quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza. Dobbiamo porre fine alla stagione dell'emergenza infinita che ha scatenato una vera e propria «fuga dal Parlamento», all'interno di una cornice di crisi di legittimità che stanno vivendo le istituzioni italiane e i partiti, una crisi che si affianca alla crisi economica e a una più ampia crisi della politica. Il momento eccezionale ha suscitato una reazione incredibile del sistema istituzionale: la novità assoluta della rielezione di Giorgio Napolitano non poteva non essere costituzionalmente e doverosamente necessaria per rispondere ad un momento, appunto, di crisi della politica, che ha visto l'affermarsi del «partito dell'astensione» come primo partito. Questa crisi della politica non deve trasformarsi in una crisi delle politiche. Non possiamo più permettere che il Parlamento sia messo in secondo piano nel momento decisionale: a questo devono aiutarci le riforme costituzionali. L'articolo 5 della Costituzione riconosce le autonomie territoriali - quelle «forze vive» nella visione di Mortati - e le promuove: a questo dobbiamo mirare quando pensiamo alla riforma del bicameralismo. Una considerazione finale va fatta, allora, quanto agli strumenti partecipativi nella formazione della volontà politica e amministrativa. Condivido pienamente la necessità di una maggiore attenzione a tali strumenti. Non si pensi, però, neanche un attimo, che il ricorso alle forme partecipative ci alleggerisca del peso delle scelte; chi, come me, crede nel valore dei partiti, non può che pensare alla politica come abilità di trovare soluzioni e intese, superando le faziosità e l'incomunicabilità. Considero altresì importante dare maggiore importanza alle Regioni e ai Comuni, dando per superate le Province come da disegno di legge costituzionale il cui testo è stato già redatto. Penso alla Camera delle autonomie, perché uno Stato che non voglia avere una visione accentratrice deve dare maggior valore agli enti locali, in quanto istituzioni più vicine ai cittadini. Spesso, e in modo assolutamente improprio, i Comuni vengono individuati come i maggiori centri di spesa, i principali destinatari della scure che si deve abbattere sulla spesa pubblica, dimenticando che sono quei Comuni e i loro amministratori a soffrire dei maggiori sacrifici, anche se le necessità di dare delle risposte ai cittadini non sono rimaste inalterate, ma sono grandemente cresciute. Bene, quindi, se l'intento vuol essere quello di dare maggiore rilievo alle autonomie, principali articolazioni del nostro Stato, soprattutto se la lente di ingrandimento deve essere posta, prima di tutto, sulle strutture centrali che non mi consta essere state mai toccate, quasi si possa perseguire un intento di autoconservazione ormai non più giustificabile. Si è parlato molto di costi della politica e troppo poco dei costi della burocrazia, dei costi dell'amministrazione, delle società partecipate e di tutte le realtà che rappresentano una forte componente della spesa pubblica, ma non sono mai oggetto di esame e, conseguentemente, di critica. Signor Presidente, signor Ministro, il primo passo di oggi è importante, ma il cammino che ci attende non è facile; va quindi affrontato con decisione e con la consapevolezza che i cittadini ci hanno chiesto un cambiamento radicale, non solo una discontinuità nella guida di un Governo. La sfida con oggi è iniziata; definiamo le regole e i tempi. Credo che ormai non ci sia più spazio per i veti e per gli alibi, perché questo percorso richiede un'assoluta serietà. È un impegno che dobbiamo assumerci nei confronti del Presidente della Repubblica e soprattutto nei confronti di chi il Presidente della Repubblica rappresenta, cioè l'intero popolo italiano. Presidente, la prima considerazione che ci viene da fare è perché si procede con un disegno di legge costituzionale per svolgere attività che sono già regolate dalle vigenti disposizioni e sono nella disponibilità piena del Parlamento, sia nei tempi che nei modi. nei modi. Si pratica questa strada, ancora una volta, per fare fumo, per confondere le idee, per nascondere il vero; e siccome una delle ragioni della crisi della politica è questo modo di comportarsi, questo vizio, cioè, di dire una cosa e pensarne un'altra, il risultato che si punta ad ottenere con questo processo sarà esattamente il

di operazioni di riforma costituzionale ne incontreremmo molte, e molte riuscite. Il Titolo V della Costituzione è stato modificato

autorevolissimi rappresentanti dei partiti dell'attuale maggioranza. Si è toccata tutta la Parte II della Costituzione.

cioè, che questo Parlamento, in questi anni abbia prevalentemente fatto esattamente quello che si propone ancora di fare. È come un'ostinazione alla quale bisogna necessariamente rispondere. Noi all'apertura di ogni legislatura incominciamo a fare che cosa? La riforma della Parte II della Costituzione. È un compito: ci sarà qualche maestro da qualche parte che ce lo assegnerà puntualmente all'inizio di ogni legislatura, con esiti pessimi dal punto di vista del risultato, perché disorientiamo tutti. In tutti i documenti di cui si è discusso in questi giorni, nelle mozioni, anche quelle presentate dalla mia parte politica, anche nell'altro ramo del Parlamento, per esempio, si è passati dal federalismo spinto ‑ lo dico ai colleghi della Lega alla supremazia del Parlamento in tema di legislazione concorrente. Eppure eravate voi, quelli che c'erano in questo Parlamento, a dire che bisognava avvicinarsi al cittadino; che i territori dovevano essere partecipi e anzi protagonisti del processo di formazione delle norme; che i cittadini dovevano partecipare e scegliere più direttamente. E adesso parliamo della supremazia, nella legislazione concorrente, del Parlamento rispetto ai Consigli regionali. Anzi, pensiamo addirittura di chiuderli. Le Province vanno cancellate. E chissà cosa deve succedere dei Comuni. Abbiamo impostato tutta la materia fiscale in funzione del federalismo, e l'abbiamo fatto ieri, non l'abbiamo fatto trenta o quaranta anni fa: l'abbiamo fatto ieri! E oggi tutto quello che si combina, si combina verso una nuova forma di centralismo, anche autoritario. Bisogna infatti decidere; e decidere non bene o male: decidere diventa l'imperativo. Poi, si può decidere male: Voglio dire che questo provvedimento, al di là di essere più o meno accettabile sotto il profilo giuridico-costituzionale è veramente inaccettabile sotto il profilo politico, perché non è una risposta al bisogno dei cittadini, ma è un affronto a quel bisogno. Ed è un affronto perché i cittadini chiedono esattamente il contrario alla politica,

I cittadini criticano la politica perché si chiude. Criticano la politica perché non favorisce la partecipazione. Criticano la politica perché delude sul piano delle risposte al bisogno della comunità. Criticano la politica perché è spendacciona e perché acquisisce privilegi che consuma a suo esclusivo beneficio. Criticano la politica perché costruisce attorno a sé una roccaforte di difesa, forse neppure del privilegio personale, ma comunque della sua funzione di potere anche quando questo potere diventa un esercizio inutile. Rispetto a queste critiche, noi facciamo una operazione di restringimento del perimetro della decisione; la proposta che viene fatta, cioè, realizza esattamente questo: circoscrive ancora di più il perimetro della partecipazione alla decisione. Intanto, quaranta parlamentari; intanto quelli che hanno certe caratteristiche; intanto, con una possibilità di intervento sulla realizzazione del progetto di legge finale, della disposizione che verrà votata e che verrà anche - come

si diano a tutti i cittadini gli identici strumenti di valutazione e di critica per consentire di esprimersi sul contenuto della proposta di legge. Tutto ciò - badate - è non solo un aggravio di fatica per questo Parlamento che dovrebbe essere impegnato a risolvere i veri problemi: come sbarcare il lunario; come riuscire ad aiutare i cittadini in maggiore difficoltà e più colpiti dalla crisi

dello sviluppo di questo Paese, di sbloccare questo Paese, di toglierlo dalla condizione nella quale si va cacciando della gestione del declino. E invece no: stabiliamo addirittura che l'attività parlamentare è residuale e che i grandi stanno tutti lì, giorno e notte, e possono anche assentarsi dall'attività ordinaria del Parlamento, quella di maggior rilievo, quella più importante, quella che risponde alla quotidianità del bisogno dei cittadini. bicamerali ne abbiamo fatte altre. Non voglio dire che fine ha fatto una famosa bicamerale e come sono cambiate le opinioni nel corso dei suoi lavori. Ma possiamo, signor Presidente, colleghi, pensare che, anche se questo lavoro fosse fatto, esso fosse fatto, esso venga fatto rispettando almeno il Parlamento, che origina questo prodotto come dire - ristretto di valutazione e di redazione di possibili sbocchi normativi di riforma costituzionale? Possiamo farlo, questo? E attenzione, perché la nostra Costituzione è un corpo armonico di norme e i principi fondamentali non sono separati dalla Parte II della Costituzione. all'articolo 5, che si devono promuovere le autonomie e diciamo anche che la legislazione e lo Stato si adeguano a quel percorso e a quel progetto di sviluppo delle autonomie, non possiamo, nella Parte II, dire l'esatto contrario. E nel fare questo progetto di legge, nel presentarlo, nel rappresentarlo all'esterno, noi stiamo pensando esattamente di fare il contrario di quello che c'è scritto nell'articolo 5 della Costituzione. Signor Presidente, io so già come finiranno le votazioni. Però sono anche molto fiducioso sul fatto che i fallimenti di questi percorsi di riforma costituzionale, veramente un po' isterici, sono sempre stati degli ottimi salvagente della nostra Costituzione.

sottoponendo un testo a questa Assemblea, la Commissione ha compiuto il primo passo di quel cammino delle riforme che costituisce uno degli obiettivi che si prefigge il Governo e con esso la maggioranza che lo sostiene. E non nascondo che questo primo passo ha suscitato in me sentimenti talora contrastanti. Sentimenti che, pur nel loro contrasto, confermano l'idea che ho espresso in Commissione e che ribadisco qui: riforme all'assetto istituzionale sono necessarie al Paese. Sono necessarie per motivi diversi: culturali, sociali, politici ed economici. Quindi, non possiamo permetterci di interrompere quel cammino; sarebbe un fallimento, non solo della maggioranza, ma di tutti. Questo è il motivo che sta alla base del consenso espresso dal mio partito alla proposta di una procedura per così dire straordinaria di revisione costituzionale. Sono soddisfatta anche per il clima e la modalità che hanno segnato i lavori della Commissione. Le polemiche, forse ineludibili, che hanno accompagnato l'emanazione del provvedimento governativo hanno lasciato il posto ad una sostanziale volontà di trovare una condivisione tra diverse e legittime letture della realtà ed aspettative di cambiamento della realtà stessa. Mi sembra che sia stato proprio questo clima a consentire il superamento, ad esempio, di alcune perplessità di ordine tecnico che avevo anche sottoposto all'attenzione dei colleghi nel corso della discussione: penso alle modifiche intervenute che hanno portato a chiarire come l'elemento tempestività del provvedimento non possa far premio sulla funzione del Parlamento. Ciò avrebbe rischiato di far superare il confine tra le prerogative costituzionalmente segnate degli organi legislativo ed esecutivo. Bene, dunque, la correzione apportata all'organizzazione dei lavori, che consente al Parlamento di valutare l'opportunità di avere a disposizione tempi più ragionevoli per concludere i propri lavori. modo, non posso non salutare favorevolmente la ridefinizione, o meglio la semplificazione, delle modalità operative attribuite all'originario Sottocomitato che funge da relatore nei lavori nelle Assemblee delle due Camere. Nell'originario testo, quelle modalità risultavano effettivamente macchinose e lasciavano impregiudicato il dubbio se la prevista partecipazione collegiale potesse influire o meno sulla formazione delle maggioranze nelle Assemblee e quale dovesse essere eventualmente il rimedio. Ma l'aspetto più rilevante credo possa individuarsi nell'aver trovato una soluzione ad una questione per la quale rischiavamo *l'impasse*: quella che può definirsi l'oggetto dei lavori del Comitato parlamentare. L'intesa intervenuta ha portato all'emendamento all'articolo 2 della relatrice, la presidente Finocchiaro, che ha consentito di razionalizzare la precedente formulazione, sanando alcune incertezze, come, ad esempio, il significato della coerenza che il di segno di legge originario prescriveva per i progetti di riforma riforma dei diversi titoli e i relativi sistemi elettorali. Ma qui gli aspetti positivi lasciano il posto all'amarezza. Tralascerei le perplessità che permangono, relative al rapporto il gruppo di 35 esperti di cui il Governo intende avvalersi, come scritto nella mozione di indirizzo approvata. Mi concentrerei piuttosto su un aspetto rilevante dell'emendamento della presidente Finocchiaro, prodotto, come dicevo poco fa, di un'intesa, ma soprattutto di una precedente tensione, legato alla possibilità di introdurre anche il Titolo IV tra quelli oggetto della revisione. Questa possibile introduzione è stata vista come uno strappo, aggettivato peraltro come inaccettabile da persone che addirittura si sono fatte paladine della giustizia tanto da affermare che essa, come si leggeva sui giornali di qualche giorno fa, «non può essere il terreno su cui scaricare vicende estranee agli obiettivi di riforma e ammodernamento dell'assetto istituzionale». Non siamo di fronte ad un politico strappo o, addirittura, ad un più marziale *blitz*. Su questo penso ci sia stata un'incomprensione. Tirare dentro la discussione anche del Titolo IV, quello sulla magistratura, ha un significato prettamente tecnico. Mi chiedo: come si fa a voler riformare Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Regioni, Province e Comuni, saltando a piè pari il Titolo IV? È certamente superfluo ricordare, ad esempio, che il Presidente della Repubblica è anche Presidente del CSM. modo mi sembra evidente che se il Parlamento decidesse per un qualsiasi sistema presidenziale sarà pure necessario esaminare e valutare quali risvolti ci sarebbero nel rapporto tra un organo e un ordine dello Stato. E, se il Senato, poi dovesse diventare una Camera delle Regioni, potrebbe vantare il diritto di nomina di componenti la Corte costituzionale? Non ci sarebbe la necessità di verificare anche qui l'eventuale modalità di nomina? La mia amarezza sta nel fatto che dietro quelle affermazioni, al presunto *blitz*, si celano pregiudizi, profondi e perduranti, che si manifestano ogni volta che si tocca la questione giustizia, che è volutamente mantenuta connessa a Silvio Berlusconi. Ma quale sarebbe il nesso tra l'emendamento incriminato e Berlusconi? Si tratta, però, di un pregiudizio che impedisce di affrontare adeguatamente ed in tutta la sua portata un aspetto cruciale della vita presente e soprattutto futura del Paese. Riusciamo solo ad affrontarlo con un atteggiamento ipocrita e per certi versi sconsiderato! Mi sembra superfluo ricordare come emerga chiaramente dal Paese l'urgenza di una riforma di un settore centrale della vita istituzionale. Tutti - e ormai non più solo qualcuno - continuano a dire che la giustizia è ormai diventata un'emergenza sociale ed economica. Basti ricordare qualche dato: il sovraffollamento carcerario è oggetto di provvedimenti di necessità e di urgenza; il presidente dell'ENI ricordava, qualche giorno fa, che siamo al 45° posto nel mondo per attrattività e che le multinazionali per investire chiedono interventi efficaci sulla giustizia, un'urgenza che la Banca mondiale ci ricorda ancora una volta nel Doing Business 2013. Ma tutto ciò, purtroppo, diventa secondario rispetto all'ossessione Berlusconi. L'invito a questa Assemblea è, quindi, duplice. Innanzitutto, solo in questo modo sarà possibile evitare il rischio di impelagarsi in polemiche su argomenti limitrofi, come ad esempio il destino del "porcellum" e le possibili alternative elettorali. affrontare con atteggiamento laico un compito che non possiamo ulteriormente procrastinare. In caso contrario, come dicevo all'inizio, perderemmo tutti.

che, rispetto a quegli argomenti concernenti i tanti insuccessi degli ultimi trent'anni, dalla Commissione Bozzi a oggi, nella relazione della collega Finocchiaro non si sia adeguatamente focalizzato quando invece riforme della Costituzione improvvisate, improvvide e faziose hanno avuto successo, e quanto male hanno recato al nostro ordinamento. Mi riferisco - e procedo per *flashback* alla riforma del 2001, quella del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha reso francamente ridicolo e imbarazzante in Europa Ma come si fa a parlare di quella riforma, senza guardare alla legislazione ordinaria che con tanta superficialità e con tanto cinismo l'aveva preceduta? Sto parlando delle cosiddette leggi Bassanini: eravamo nella seconda metà degli anni Novanta, veniva preso a picconate lo Stato, e ci si vantava di fare le riforme a Costituzione invariata. Una destra tutt'altro che lungimirante, faziosa e pasticciona, i Feltri e i Montanelli benedivano le leggi Bassanini con lo stesso cinismo con il quale qualche anno fa Rizzo Rizzo e Stella sono diventati cattedratici di costituzionalismo quasi quotidiano. Quella riforma nacque dalla faziosità dei colleghi della sinistra che, per rappresaglia nei confronti dei colleghi della Lega che stavano per scegliere l'alleanza con il centrodestra, regalarono loro quel bel tipo di federalismo. Questo quadro costituzionale è un'emergenza nella quale ci incartiamo giorno per giorno. Non è soltanto il senatore Gasparri a polemizzare con l'attuale Ministro dell'economia: la polemica fra il Parlamento e il Ministro dell'economia risale proprio al qualunquistico obbrobrio delle leggi Bassanini. Ma vi rendete conto che Palazzo Chigi è una bicicletta e che il Ministero dell'economia è più di un carro armato? E vi rendete conto che l'istituzione costituzionale del Governo in Parlamento, a prescindere dalle questioni personali (Saccomanni, Tremonti, Padoa-Schioppa),

con tantissima improvvisazione, tant'è vero che quando noi varammo le Regioni le definimmo organi di legislazione e di programmazione, ma mai di gestione? Che fu il 1970? Localismo cinico e e fascista nel senso peggiore. Io facevo il soldato, dovevo tenere l'ordine pubblico a Reggio Calabria, dove si alternavano Ciccio Franco, Adriano Sofri ed Amedeo Matacena: che bell'inizio! In Abruzzo fu ancora peggio: Pescara contro L'Aquila e L'Aquila contro Pescara. In Campania si decise di astenersi per una legislatura intera. La lotta fra zone costiere e zone interne, De Mita contro Gava, non era arbitrabile neanche dalla consueta giunta Leone (Carlo Leone),

Le Regioni come sportello, le Regioni come comune in grande, le Regioni come gestione. Signor Ministro, conosco la drammatica scadenza della questione delle Province, ma siamo intellettualmente onesti: l'abrogazione delle Province aveva un senso in quell'epoca, quando in piazza scendevano Sofri e Ciccio Franco e il Governo Colombo prometteva il quinto sito siderurgico a Gioia Tauro. Che bella pensata! Oggi la corsa alle Province è stata com'era stata prima di allora, si vuole l'istituzione Provincia perché si vuole lo Stato, si vuole il provveditore agli studi, si vuole il provveditore alle opere pubbliche, tutto quello che le leggi Bassanini hanno abrogato. Non c'è più lo Stato. Per quanto abilissima sia una collega come la senatrice nel lessico costituente-costituito, il lessico della Costituzione attuale ha cancellato lo Stato: lo Stato segue le Regioni e le altre autonomie, e persino le comunità montane. Il riferimento unitario della Repubblica non è più lo Stato: cioè, è stato picconato ed ucciso il riferimento di modernità con il quale nel 1860 nacque lo lo Stato nazionale. Quanto allo Stato in periferia, sono restate soltanto le soprintendenze ai beni culturali, svuotate di poteri e di denaro rispetto alle Regioni, perché la contingenza volle che il Ministro del settore, l'onorevole Veltroni, fosse Vice Presidente del Consiglio, e volle strappare questa coccarda al collega riformatore Bassanini. E allora come si fa, senatori o deputati che si sia, ad auspicare che un glorioso ramo del nostro Parlamento diventi una sorta di Conferenza Stato-Regioni? Ma voi ci siete mai stati in Conferenza Stato-Regioni? Una compagnia dialettale, nell'accezione più benevola. Ma voi siete mai stati in Germania, a dire che loro hanno i *Länder* e noi abbiamo le Regioni? Fino a qualche anno fa si mettevano a ridere, oggi dicono: non ci offendete. E la storia dei nostri fallimenti in Europa, dell'Italia in Europa e dell'Europa in Italia, deve tutto o per lo meno quasi tutto al nostro regionalismo scombiccherato. Veniamo all'attualità, all'emergenza: tagliare la spesa pubblica con questo ordinamento costituzionale è diventato impossibile. L'ultima volta che ci riuscimmo in modo significativo era al principio degli anni Novanta. Governo c'era Amato, ingenerosamente rubricato come il Presidente del Consiglio che mise le mani nelle tasche degli italiani, il che fece;

al Governo, quella sul pubblico impiego; una era sulle pensioni, un'altra sulla sanità e l'ultima sulla finanza territoriale. Oggi tutto questo è proibito dalla Costituzione. La nostra evocazione di tagli alla spesa pubblica è affidata al nulla. E allora, signor Ministro, stiamo molto attenti. Eravamo insieme sugli stessi banchi, e il nostro presidente di Gruppo era il senatore Gasparri, il tema delle Province fu introdotto dal Governo Monti in modo disordinato e fazioso, quasi a voler tacere su quello che era il malato il malato canceroso, e con le metastasi: la finanza regionale. Stiamo attenti, nelle prossime settimane ci occuperemo di questo aspetto. critico il qualunquismo indotto da Rizzo e Stella, però io Rizzo e Stella li leggo, e mi ha fatto male come cittadino italiano

bello, infatti, è che c'è un regionalismo che per i primi dieci anni non voleva essere ente locale; oggi, invece, le Regioni rivendicano ancora più localismo degli enti locali: moltiplicazioni di competenze, sovrapposizione di funzioni, sprechi ineliminabili, assumere senza concorso né incappare nel divieto del *turnover*. Soltanto nel 2008, cioè cinque anni fa, la Corte dei conti, che pure non ci può fare niente in questo baobab delle società partecipate, calcolava che questa massa informe di imprese pubbliche (la parola imprese non la mettevano fra virgolette: forse non era colpa loro) occupi 255.000 persone, oltre a 38.000 fra consiglieri di amministrazione, revisori contabili e alti dirigenti. E poi si vuole far credere che l'oggetto delle riforme costituzionali debba essere il numero dei parlamentari! Questo è qualunquismo e insieme cinismo. L'altra riforma costituzionale che purtroppo ha avuto successo nella storia del nostro sfortunato Paese fu quella che la collega Alberti Casellati chiamerebbe «della giustizia». Io non la chiamo così, perché anche quando riguarda la giurisdizione, ciò che è costituzionale è un solo tema: la libertà e le garanzie della libertà. Nel 1993 una piazza fascista, nel senso deteriore, impose al libero Parlamento italiano una modifica dell'articolo 68 della Costituzione che grida ancora vergogna. Il Senato votò un proprio testo; lo propose un collega di cui avevo grandissima stima: il collega Maccanico. Questo testo non ha mai potuto essere esaminato alla Camera dei deputati, seppellito sotto gli squadristi che buttavano le monetine contro Craxi, anche in quel caso dopo un libero voto della Camera dei deputati, opinabile quanto si vuole, ma non certo per le condizioni di libertà nelle quali era stato espresso. Che cosa è la sfida della giustizia contro la politica se non l'abbattimento di quelle garanzie dell'articolo 68? Del resto - qualche amico della Commissione giustizia lo ricorderà - quando dieci anni prima si era modificato il codice di procedura penale (era stato un grande momento di Pisapia padre), si era detto: sì, questo questo va bene, ma se non arriva subito in Costituzione e nell'ordinamento la divisione delle carriere, la divisione dei profili fra chi accusa e chi giudica, sarà un biliardino che fa *tilt*. E così accadde. E così accadde anche durante il tentativo che sembrò andare a buon fine (c'era una Bicamerale presieduta da D'Alema) a casa di Letta (qui Giuliano Ferrara direbbe: inteso come "il conte zio" e non come il Presidente del Consiglio): si fece un accordo sulla materia elettorale, estranea o comunque laterale alla Costituzione. Fu definito il "patto della crostata". Nei giorni successivi ci si accorse che, per quanto il patto della crostata fosse solido, c'era un cittadino italiano al quale veniva propinato come pietanza il risotto alla milanese, e soltanto quello. Ci fu un Presidente della Repubblica che disonorò la sua funzione aggredendo il Parlamento. Quando la Bicamerale doveva portare all'attenzione dell'Aula i propri lavori, mandò un telegramma ad un congresso di magistrati dicendo che mai avrebbe promulgato una legge che avesse distinto i profili all'interno della magistratura. Perché fu sconsiderato quel messaggio? Perché in quel Parlamento c'era ben il 50 per cento di disegni di legge in questo senso. E siccome io rispetto il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, il Presidente della Repubblica forse sbagliò, ma esercitò il suo diritto‑dovere. Quello che fu veramente agghiacciante ed assordante fu il silenzio del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Vedete, colleghi, fra i valori costituzionali c'è certamente quello che più volte viene ripetuto da dieci anni come un bla bla bla: indipendenza ed autonomia della magistratura. Malgrado quel che si può pensare, quel valore lo rispetto anche io, però rispetto altrettanto l'indipendenza e l'autonomia dalla magistratura. Quella sconsiderata riforma dell'articolo 68 della Costituzione ci ha privato di risorse di indipendenza e di autonomia dalla magistratura

da aggressioni populistiche, da intimazioni accademiche dei consigli di facoltà la centralità del Parlamento, avesse avuto anche nel suo animo implicito quel valore di indipendenza e di autonomia dalla magistratura che è nella storia di queste istituzioni e nella storia d'Italia. Colleghi della sinistra, vi siete mai domandati per quali ragioni nel '48, nel '53, nel '58 e nel '63 la maggioranza anticomunista votasse senza esitazione il rifiuto all'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Moranino? Il problema lo risolse Saragat nel 1964 con la grazia. Non lo facevamo perché il nostro anticomunismo era disposto a venire a patti, ma in nome di un valore antico che è sempre moderno, quello con il quale mi piace concludere oggi, ricordando a me stesso e a voi tutti l'altro ieri sui giornali c'era una bella notizia: l'ex collega Tedesco è stato prosciolto. Pertanto, quell'idea di una politica sottoposta a processo popolare, evocata prima da un collega,

per l'ennesima volta in vent'anni nella Seconda Repubblica si apre una discussione su riforme istituzionali da consacrare in apposite ed esplicite riforme costituzionali. Questa volta la discussione dovrebbe essere avvantaggiata dai numeri del Governo delle larghe intese (in Parlamento, ma non nel Paese). Nei dibattiti che hanno preceduto in queste settimane il disegno di legge costituzionale, tutti i colleghi della maggioranza hanno ampiamente sostenuto che non è in atto nessuna riforma costituzionale fuori dai principi della Carta del 1948 e che, soprattutto, questa riforma non dovrà mai disegnare una nuova forma di Stato, come stamani la presidente Finocchiario ha ribadito, né un sistema presidenziale, né semipresidenziale sul modello francese. Toni solenni si sono sollevati in quest'Aula e nel Paese da esponenti autorevoli della maggioranza a difesa del nostro sistema repubblicano e parlamentare. ecco che tutti si sono autosmentiti alla prima prova, perché, come abbiamo sostenuto nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, siamo dinanzi ad una palese violazione dell'articolo 71, dell'articolo 72 e dell'articolo 138 Articolo 138 non rispettato persino nel dimezzamento della pausa di riflessione, previsto dall'articolo 4 di questo disegno di legge, in evidente contrasto con la Carta del 1948, che prevede che la pausa non possa essere inferiore a tre mesi. Questa scelta venne fatta per permettere alle eventuali riforme costituzionali di essere adeguatamente discusse nell'opinione pubblica in un aperto confronto con il dibattito parlamentare. In questi ultimi vent'anni abbiamo già assistito a due riforme costituzionali, approvate sempre a maggioranza, per la scelta chiara di non ricercare il più ampio consenso politicamente trasversale in Parlamento. L'una, seppure avallata da un *referendum*, viene oggi criticata perfino da alcuni tra coloro che la appoggiarono e sostennero a quel tempo, votata in quel caso dal solo centrosinistra. L'ultima, avanzata dal centrodestra, è stata bocciata da un *referendum* popolare che ha detto no ad un più che evidente segno presidenzialista. In questi anni, abbiamo visto tre volte cambiare la legge elettorale: dal sistema proporzionale che ci ha accompagnato dall'inizio della nostra Repubblica ad un sistema con collegi maggioritari e una parte proporzionale, sostituito con il "porcellum" che, nelle peggiori tradizioni della dittatura della maggioranza, è un modello che aveva come obiettivo l'instabilità elettorale al Senato, con un meccanismo che oggi è posto sotto osservazione anche per dubbia costituzionalità. Nel disegno di legge è scritto che saranno esaminate dal Comitato leggi elettorali solo se conseguenti alla revisione della Costituzione. Nulla vieta alle Commissioni referenti di lavorare su una nuova legge elettorale, necessaria per restituire quel diritto di scelta e partecipazione ai cittadini negato totalmente dal "porcellum". Peccato che la maggioranza abbia fatto altra scelta, come confermano le parole del Presidente della Repubblica

ha sostenuto sempre la presidente Finocchiario. Per noi, lo abbiamo detto più volte, il tema dovrebbe essere la piena attuazione della Costituzione e l'effettiva operatività di tutti diritti. Di fronte a questi tentativi di cambiare la nostra architettura costituzionale ed elettorale, abbiamo visto variare maggioranze parlamentari, a volte anche estese, che non sempre sono riuscite a rendere effettive le scelte di Governo. Dal 1983, con la prima Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, si prova a cambiare questa architettura, con risultati a volte nefasti o controproducenti, come tanti interventi hanno sottolineato. Se guardiamo bene, l'unica riforma che abbia avuto un certo grado di efficienza è quella del sistema elettorale ed istituzionale dei Comuni, che dà garanzia di governabilità mantenendo un certo grado di pluralismo, pur con tutte le criticità per il forte rischio di svuotamento del ruolo delle assemblee elettive e forti poteri concentrati nella figura del sindaco. È una legge che avete modificato nella scorsa legislatura solo per ridurre gli spazi di rappresentanza e di democrazia. In questo dibattito è stato evocato più volte il tema della governabilità, che è diventato in un certo senso un *totem* ed un alibi al tempo stesso. Noi siamo stati eletti in Parlamento, senza vincolo di mandato imperativo, per rappresentare il popolo italiano. Tuttavia ad ogni elezione crolla sempre di più il numero degli elettori; questo significa che il popolo si riconosce sempre meno nei suoi eletti. Certo, i casi di corruzione, contiguità alla criminalità organizzata, malaffare, gestione scorretta dei finanziamenti pubblici ai partiti non hanno aiutato. I cittadini vogliono essere rappresentati da persone di cui condividono progetti, aspettative, ideali e interessi legittimi. Vedere invece grandi coalizioni di Governo immobili, che delegano la politica a tecnici, sia che vengano dall'Europa o da fondazioni simil-universitarie legate a partiti o ad esponenti politici, allontana la voglia di partecipazione. In nome della governabilità si pensa di dover fare una riforma costituzionale, ma questo non farà scomparire le forti contraddizioni presenti in alcune forze politiche, come abbiamo avuto occasione di vedere durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Non basterà la vostra riforma a riavvicinare i cittadini alla politica. La governabilità è diventata un *totem* perché non sempre bastano i grandi numeri per governare, come abbiamo visto nella passata legislatura dove l'incredibile maggioranza che sosteneva il Governo di centrodestra non è bastata. La governabilità è anche un alibi perché, se non bastano i numeri per governare, la si usa come scusa per cancellare la rappresentazione della società politica dal Parlamento. Cambiare la Costituzione con l'imposizione della maggioranza, cercando maldestramente di spiegare ai cittadini l'ineluttabilità della scelta in nome di quel *totem* e di quell'alibi, affidare ai saggi la guida di questo importante processo di cambiamento: sarà tutto inutile se non ritorna la politica, se non ritorna la condivisione di ideali e di valori. Nessun saggio, nessuna riforma, nessuna legge elettorale supplirà alla carenza di politica, alla carenza di idee e di libero confronto. Non siamo oggi nell'immediato dopoguerra, dopo il fascismo, non siamo agli albori della democrazia italiana. La Costituzione fu comunque decisa dai costituenti eletti in modo proporzionale e con il coinvolgimento di quasi tutte le forze politiche politiche democratiche. Lì c'era da ricostruire un Paese e si presero due anni. Qui dobbiamo lasciarci alle spalle gli scandali, la mala politica dei furbi e vogliamo fare una rivoluzione copernicana in tre mesi. Forse stiamo superando ogni limite. Affrontare con coerenza i problemi ci consentirà di superare questa fase di crisi culturale e morale della politica, recuperando non solo la dignità delle istituzioni, attraverso la trasparenza e l'etica, ma anche la forza dell'azione politica. Questa maggioranza delle larghe intese è davvero singolare: ha difficoltà a trovare unità di intenti sull'IMU o sull'aumento dell'IVA - e ne capiamo le ragioni, perché dovrebbe trattarsi di due idee diverse di sviluppo ma trova una strana coesione su un atto che mette seriamente in discussione l'essenza della Repubblica democratica. In questo processo di riforma per noi c'è solo il brutto tentativo di cancellare la politica, quella vera, e la partecipazione di tutti i cittadini in un goffo tentativo di autoconservazione.

sono passati quasi vent'anni da quando si iniziò ad avvertire l'esigenza di rinnovare e riformare il sistema Paese attraverso le necessarie modifiche costituzionali: un'esigenza largamente condivisa, che trovava la sua forza ispiratrice dal basso, dalle attese e delle aspettative avvertite dai cittadini, dalla società civile. La società aveva iniziato a prendere consapevolezza del fatto che il nuovo assetto mondiale ed europeo presupponesse modifiche strutturali capaci di ridisegnare l'organizzazione dello Stato in modo più dinamico e funzionale. Questa necessità di cambiamento ha però, nei fatti, incontrato ostacoli insormontabili e si è dovuta scontrare con le posizioni ortodosse, miopi ed ideologiche degli "ultras" della teoria dell'intangibilità della Costituzione. Ricordiamo tutti i paladini di questa pseudovisione precostituita che ha elevato la Costituzione a verbo incarnato manifestare il proprio dissenso contro qualsiasi volontà di cambiamento. Le suggestive motivazioni che venivano e vengono addotte a suffragio della sacralità della Carta costituzionale sono fondate, giustamente, sul rispetto del lavoro encomiabile che fu condotto dai Padri costituenti nel dopoguerra quale sintesi del pensiero delle diverse anime che avevano contribuito a far uscire il nostro Paese dalla dittatura fascista. Lungi da me non comprendere e non sottolineare l'importanza storica (e non solo) che incarna la Carta fondamentale, in particolar modo nei suoi primi articoli che enunciano i principi fondamentali sui quali si fonda la nostra democrazia nelle sue declinazioni di rispetto dell'uguaglianza tra i cittadini, dei diritti e delle libertà personali inviolabili. Le posizioni ideologiche, conservatrici e di retroguardia, però, hanno prodotto negli anni uno spaventoso immobilismo che ha infettato pian piano tutte le strutture del sistema statale. Questa latente, diffusa, soporifera inerzia ha indebolito il nostro Paese, ponendolo al rischio di una irreversibile malattia. L'ipocrisia e va sottolineato - di certi atteggiamenti conservatori e anacronistici non ha permesso in tutti questi anni di addivenire ad una modifica sostanziale dell'assetto organizzativo di questo Stato, capace realmente di andare ad incidere in modo preponderante nel sistema, ridisegnandolo fin dalle sue fondamenta e rendendolo finalmente capace nella sua nuova struttura di affrontare i cambiamenti della società in modo tale da presentarlo, da protagonista, nel nuovo contesto internazionale internazionale ed europeo. Nella storia di uno Stato, qualora non si sia capaci con lungimiranza di adottare nei tempi giusti le necessarie riforme attraverso una programmazione di lungo periodo,

intervengono degli eventi drammatici, dei fattori scatenanti che sconvolgono gli assetti e che, se non governati, possono irrimediabilmente causare degli stravolgimenti tali che per la loro portata rischiano di non essere indolori. La congiuntura economica internazionale che ha investito il mondo e che ha avuto pesanti ripercussioni anche nel nostro Paese ha fatto emergere tutti i mali di un sistema immobile affetto da una burocrazia elefantiaca, incapace di responsabilizzare gli amministratori, sempre più distante dalle necessità reali dei un sistema improduttivo e assistenzialista inadeguato alla valorizzazione dei territori, organizzato senza alcun rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, fagocitato da una politica autoreferenziale dimentica del suo primario suo primario compito di ricerca del bene comune, ma basata esclusivamente sul consenso elettorale. Quello che in tutti questi anni doveva essere fatto e non è stato fatto è oggi improcrastinabile. Non è il Governo, non siamo noi parlamentari a condurre questa fase di riforme, colleghi: è il popolo che le vuole, che le ha chieste con forza come ultimo appello alla politica. O la politica sarà capace di cambiare e rinnovarsi o non ci sarà data una seconda possibilità. Spiace, peraltro, constatare che tra i banchi delle forze politiche che sostengono il Governo vi è il vuoto, vi sono

esclusivamente per attenuare l'energia prorompente della Lega Nord, che sempre più si radicava quale forza di impatto per far emergere la questione settentrionale completamente sottovalutata. I giochi di palazzo orchestrati ad arte per rallentare quelle riforme che andavano direttamente ad incidere sugli interessi degli apparati statali e di palazzo oggi non sono più accettabili. Cosa dire poi delle campagne ideologiche che sono state sostenute da alcune forze politiche per arrestare quelle riforme, come la cosiddetta *devolution*,

che prevedeva già l'istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei parlamentari, di cui tutti discutono, modifiche al procedimento di formazione delle leggi

dal volere veramente il federalismo e dall'agire con convinzione e determinazione per cambiare il sistema Paese, questo disegno di legge di riforma - mi riferisco alla devoluzione - fu respinto, come già detto, con il *referendum* confermativo del giugno 2006. La campagna per votare no fu manovrata ad arte da quelle stesse forze politiche che, a parole, si dichiaravano - e si dichiarano oggi - a favore del federalismo, a favore cioè dell'ammodernamento e dell'efficientamento del Paese e della responsabilizzazione finalmente nell'utilizzo delle risorse pubbliche dappertutto. Unica *chance* di riscatto del Paese, Avviandomi alle conclusioni, lasciate che ribadisca che la mia - la nostra - è la speranza di vedere oggi avviato davvero il processo di riforma, non più procrastinabile; di vedere, finalmente e concretamente, concludersi in questa legislatura il processo di riforme. È una speranza che deriva unicamente dal modo con cui si è formato questo Governo, imposto da un Presidente della Repubblica che, seppure stanco, è stato costretto ad accettare il suo secondo mandato, spinto da un senso di responsabilità e comprendendo comprendendo la straordinarietà del periodo storico che stiamo attraversando. Un Presidente che, nel momento del suo insediamento, ha ammonito i parlamentari tutti - anche quelli assenti oggi tra questi banchi - sulla necessità di giungere in tempi rapidi ad un cambiamento radicale del sistema Stato, che restituisca dignità alle istituzioni ed attenui il sentimento diffuso e comprensibile di disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni.

ha sottolineato più volte la necessità di fare tutto il possibile - e anche l'impossibile - per chiudere in tempi brevi e in modo condiviso il processo di riforma della Parte Seconda della Costituzione e la conseguente riforma elettorale, con completamento ed attuazione del percorso del federalismo fiscale. Altrimenti - è lo stesso Presidente del Consiglio ad averlo più volte ribadito - saranno assunte le conseguenti determinazioni: tutti a casa! Tutto ciò detto, auspichiamo che in questa legislatura si possa veramente riuscire ad approvare le riforme, non soltanto grazie a questi fattori straordinari, ma perché sono i cittadini, le famiglie, gli imprenditori, insomma il popolo che le vogliono e le chiedono e che faranno di tutto per ottenerle. Noi del Gruppo della Lega Nord ci siamo, perché le riforme costituzionali sono nel nostro DNA. Noi ci siamo perché, proprio grazie a noi, in questo Paese è maturata la necessità di un cambiamento essenziale: un'evoluzione profonda e di sistema. Ci siamo e abbiamo dimostrato di volere e saper dare il nostro fattivo contributo, anche in occasione dell'esame del presente disegno di legge costituzionale, con gli emendamenti migliorativi che abbiamo presentato e vari ordini del giorno, che illustreremo, di buon senso e di responsabilità. Noi siamo per un cambiamento vero, verso la modernizzazione della pubblica amministrazione, per adeguarla alle esigenze della società, per semplificare gli adempimenti e adeguare la nostra legislazione a quell'Europa più avanzata a cui tanto si fa riferimento. Siamo, soprattutto, per valorizzare le autonomie e le specificità territoriali, per la realizzazione delle macroregioni, che vengono sostenute ora finalmente anche in sede europea, per rispondere ai bisogni del mondo imprenditoriale e dei cittadini, per rendere competitivo il Paese. Non ci sono più alibi: il superamento di una visione centralista dell'architettura e dell'amministrazione statale è l'unica speranza di ripresa del Paese. *(Applausi

chiedono queste riforme istituzionali. Sinceramente, a noi non sembra che stiano bramando le riforme dell'assetto istituzionale, né il presidenzialismo, né il bicameralismo. il 16 novembre 2005 è stata approvata una nuova forma dell'assetto istituzionale, che prevedeva proprio il superamento del bicameralismo perfetto, e quella norma è stata bocciata con un *referendum*: bocciata! *(Applausi che questo termine sia costantemente nelle nostre menti: i cittadini hanno bocciato una riforma dell'assetto istituzionale nella direzione del superamento del bicameralismo perfetto. Questo è un fatto, ma noi ostinatamente continuiamo, come diceva anche il collega Uras, e perseveriamo nel cercare nuovamente di andare in direzione diversa rispetto a quello che chiedono i cittadini: lo abbiamo fatto con il nucleare, lo abbiamo fatto con i rimborsi elettorali. Ogni volta che i cittadini si esprimono, questa classe politica continua a perseverare in una strada diversa per autoproteggersi, per autotutelarsi. Si cerca un capro espiatorio; oggi si sta cercando un capro espiatorio per giustificare l'inadeguatezza di chi negli ultimi vent'anni (ma forse trenta, quaranta, cinquanta) ha governato questo Paese. Il capro espiatorio è lo strumento: siccome lo strumento non è valido,

anni chiuse nei cassetti del Senato, rimpallandole di Commissione in Commissione. Quel disegno di legge di iniziativa popolare aveva il diritto di essere portato in Aula. Oggi ci riempiamo la bocca di cittadini, di popolo, di cosa chiedono. I cittadini avevano chiesto che in quest'Aula si discutesse un disegno di legge di iniziativa popolare, e mai un provvedimento di iniziativa popolare è

in giornata. Poteva essere fatto per quei provvedimenti che hanno più diritto di stare in quest'Aula, i disegni di legge di iniziativa popolare, rispetto a quelli del Governo. Ripeto, del Governo, non del Parlamento.

Peccato fosse quello che avevamo proposto nella nostra mozione, che è stata bocciata e denigrata e che ora diventa l'iniziativa del Governo. Teniamo a precisare la nostra mozione andava proprio in tal senso. Chiedeva una grande consultazione popolare via *web* (e non solo), dopo un lungo dibattito in cui i cittadini potevano dire la loro opinione e dare un indirizzo

è ormai consueto, da 20 anni a questa parte, parlare a ogni legislatura di riforme dell'assetto istituzionale; e alla fine le riforme non si fanno. Anche in questo caso, ci rendiamo conto che questo disegno di legge costituzionale altro non

io penso che questo Parlamento sia di fronte a un bivio abbastanza serio e drammatico per il Paese, perché

o assistere impotenti allo sfascio economico e sociale di questo Paese (e ne abbiamo un esempio a pochi chilometri da noi, in Grecia)

e SEL, e alcuni a titolo personale, come il senatore Tocci, hanno detto che le riforme istituzionali non sono utili. Premetto che ho grande rispetto per tutti noi e, a maggior ragione, per i rappresentanti dell'opposizione che fanno seriamente il proprio lavoro.

che, tra la circoscrizione (o i municipi, per quanto riguarda le grandi città), il Comune, la Provincia, la Regione, la soprintendenza e il responsabile dei beni ambientali, alla fine non si sa mai chi deve decidere. Signori, non è un caso se nel nostro Paese non investono più gli stranieri; anzi, molti imprenditori italiani se ne vanno e delocalizzano. Assistiamo ad investimenti di capitali stranieri solo nel superlusso o in attività già avviate e, che non hanno bisogno di autorizzazioni o di licenze e che non hanno neanche bisogno, per come si svolgono, della giustizia ordinaria, civile. Tutti noi sappiamo infatti che, se abbiamo un credito, dobbiamo solo sperare che il nostro debitore paghi, perché, diversamente non abbiamo mezzi per perseguirlo. l'onorevole Veltroni - che ha una vasta esperienza parlamentare, che è stato Vice Presidente del Consiglio, Sindaco di una città e così via - ieri durante un dibattito televisivo ha detto una cosa vera intelligente, che rispecchia perfettamente la verità. Egli ha detto che il nostro è l'unico Paese del mondo nel quale, appena si forma un Governo, subito si parla di quello che gli deve succedere, il giorno stesso o al più tardi Questo avveniva durante la Prima Repubblica ed è continuamente avvenuto nella Seconda Repubblica, sia che le elezioni fossero state vinte dal centrodestra, sia dal centrosinistra. Abbiamo anche un caso che dimostra che quello che sto dicendo forse non è completamente sbagliato, ed è quello che avviene nei Comuni italiani. tranne in casi eccezionali, il Sindaco governa per cinque anni; magari ogni tanto cambia la Giunta, ma c'è una continuità amministrativa; alla fine i cittadini decidono se riconfermargli la fiducia, se cambiare, oppure, se ha già svolto due mandati, scegliere chi sarà il successore. Però i Comuni sono complessivamente amministrati. Noi abbiamo una macchina che è troppo lenta nel decidere, che ha competenze troppo parcellizzate e che tra l'altro, probabilmente proprio per questo, costa ai cittadini più di quanto dovrebbe costare. Nel dibattito che vi è stato oggi sono state dette cose che non mi sembra siano completamente giuste. Si è detto: si vogliono strozzare i tempi imponendoci il limite di 18 mesi. Signori, 18 mesi! Siamo in un mondo nel quale si va così in fretta che dire che 18 mesi sono pochi francamente mi sembra voler fare quasi dell'umorismo, perché non è nella realtà delle cose.

io credo che si auspichi che, attraverso la Commissione parlamentare e attraverso la consulenza di esperti, si riesca a porre il Parlamento nelle condizioni di decidere, nell'ambito di 18 mesi e con le procedure previste dall'articolo 138

non c'è dubbio che non potremo fare le riforme se non avremo la capacità di dare una risposta al dramma economico e sociale che questo Paese ha di fronte; questo è un dato di fatto.

credo che non ci saranno unanimismi e credo che ci saranno discussioni, ma penso che ne valga la pena. Io penso che, magari organizzando meglio i nostri lavori - e condivido l'opinione che una qualche revisione al nostro Regolamento Grazie,

mi sono chiesta - e lo dico con estrema sincerità - se fosse fondata l'opinione di quanti sostengono che forse bisognerebbe limitare il tempo della discussione generale, perché effettivamente spesso essa ripropone argomenti e osservazioni che dovrebbero essere maturati, verificati in Commissione; quindi questa fase può essere vissuta come una ripetizione.

e quanto è serio per noi, come dovrebbe essere per tutti, il discorso che stiamo facendo. Questo perché in Commissione non ho avuto l'impressione che stessimo perdendo tempo, e mi dispiace sentire colleghi, che in Commissione mi erano sembrati seriamente impegnati in questa discussione che, arrivati in Aula, fanno fanno propaganda (perché di questo si tratta), facile propaganda e demagogia e sostengono di perdere tempo, mentre avevano ben altri atteggiamenti quando si trattava di discutere del disegno di legge e anche dei loro emendamenti e ordini del giorno. Vorrei però iniziare il mio intervento, che sarà breve come tutti gli altri, sottolineando un dato. Noi stiamo approvando un disegno di legge che traccia un *iter* un *iter* procedurale per le riforme; lo dico perché si è parlato di tante cose in quest'Aula, giustamente, visto che chi prende la parola è libero di farlo. Spesso si è parlato anche di merito, anche se il merito non è stato proprio discusso; pertanto, anche io se parlassi di merito in questo momento esprimerei un'opinione e niente di più, perché non c'è una posizione politica da esprimere. stiamo discutendo di un *iter* procedurale che viene approvato con legge costituzionale proprio perché, a norma della Costituzione, non solo dell'articolo 138, ma anche dell'articolo 72 che qualcuno ha richiamato,

in Parlamento si vuole costituzionalizzare una procedura che non è alternativa - anzi, lavora e va nella stessa direzione - ma è leggermente diversa, sia per le leggi costituzionali che per quelle ordinarie. Pertanto, ha poco senso parlare di incostituzionalità di una legge costituzionale che, se ha un obiettivo e raggiunge un risultato è proprio quello di rendere costituzionalmente compatibili i disegni di legge che andremo ad approvare di qui in avanti, i provvedimenti che affronteranno i problemi di merito.

chiaro l'ambito della nostra discussione. Ascoltando i colleghi che sono intervenuti mi è sembrato di smarrire il senso del percorso. Si è parlato di tante cose: di travolgimenti, di fallimenti e di tante cose che evocano già risultati che noi vorremmo scongiurare. Ritorniamo però ai fatti.

con possibilità di intervenire su norme contenute in altri Titoli della Costituzione stessa, se strettamente necessario e collegato con le modifiche che vareremo.

che il Senato modifichi il proprio Regolamento: non c'è alcun ostacolo a che ciò si faccia. La stessa legge elettorale va sicuramente ed immediatamente modificata - questa almeno è la posizione del Gruppo del Partito Democratico - ma non c'è alcun ostacolo affinché ciò avvenga, e avvenga con immediatezza, e lo diciamo soprattutto

bariamo sul serio, e sappiamo che stiamo imbrogliando. Noi del Partito Democratico abbiamo condotto una campagna elettorale parlando della «Costituzione più bella del mondo» e adesso ci troveremmo invece ad essere quelli che questa Costituzione la vogliono travolgere. La verità è un'altra: i principi di quella Costituzione sono quelli che ci muovono nella direzione verso cui stiamo andando, e se c'è una differenza che oggi dobbiamo saper operare non è tra chi ama la Costituzione e chi la vuole travolgere, ma tra chi ha uno spirito innovatore e coraggioso e chi ha invece uno spirito di conservazione. Ed è strano che lo spirito di conservazione ce l'abbiano proprio

impedisce di dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione, cosa di cui in parte si sta già parlando da troppo tempo? Nessuno ci impedisce di farlo, perché la politica deve trovare un nuovo protagonismo, e lo deve fare autoregolamentandosi e varando anche anche leggi in cui sancire i propri principi. In conclusione, in questo momento dobbiamo essere assolutamente consapevoli dell'importanza della posta in gioco, e se c'è un motivo per cui mi convinco ancora di più che il Comitato è necessario è perché è necessario ed imprescindibile avere un luogo dove si parli con serietà e con serenità e dove Camera e Senato si parlino contestualmente, perché nessuna riforma si può fare se si comincia il gioco delle parti tra Camera e Senato, come è stato fatto oggi in quest'Aula maggioranza ed opposizione. Certo, mi si può dire che nel passato ci sono state tante bicamerali, eppure le riforme non si sono fatte. E allora non si tratta di di attendere il fallimento anche di questo tentativo; la domanda da porsi è perché questo è successo, quali sono i correttivi, cosa dobbiamo metterci di più in termini di passione, senso civico e senso delle istituzioni nel portare avanti queste riforme. Non si deve sempre dire di no a tutto. no a tutto. Probabilmente in questo momento il compito che noi abbiamo (non mi riferisco solo alla maggioranza, ma alla classe politica del nostro Paese) è quello di rendere credibile il nostro Paese, di renderlo competitivo sul piano istituzionale, credibile e competitivo anche sul piano economico, e tutto questo non può prescindere dalle riforme. Ricordatevi i richiami che spesso ascoltiamo quando si parla di Italia: per crederci, anche fuori dall'Italia, hanno bisogno di sapere che siamo capaci di andare oltre oltre la conservazione dell'esistente, perché quello che c'è non ci ha assicurato né la governabilità, né la capacità di decidere e di cambiare le regole del gioco quando necessario, né soprattutto, di salvare l'economia del nostro Paese. Grazie,

attengono anche a versanti che sono quelli propri della discussione sulle riforme costituzionali che ci troveremo ad affrontare.

ma di potere costituito, di modificazione di parti diverse della Costituzione, strumenti che consentissero una maggiore concentrazione e meditazione, nonché un contemperamento delle opposte posizioni

(e questo non so se sia strettamente nell'ambito della funzione del relatore, forse mi sto arrogando un diritto di parola che non avrei, ma lasciatemelo dire, colleghi), considerato che la centralità del Parlamento è stata al centro della nostra riflessione, negli interventi di tutti i colleghi, di qualunque gruppo politico, ed è stata anche la prima preoccupazione sulla base della quale siamo arrivati al testo oggi all'esame il Governo ha lasciato posizioni precedentemente delineate appunto per giungere ad un testo che celebrasse la centralità del Parlamento nell'ambito provo un certo disagio nell'ascoltare tanti giudizi in ordine alla legittimazione di quest'Aula e della Camera a decidere sulla riforma costituzionale.

alcuni colleghi hanno parlato addirittura di assenza di legittimazione morale ad affrontare questo tema. Rispetto le opinioni di tutti, che sono tutte sacre qui dentro, però credo che quando si è in quest'Aula, visto che ci si è perché si è fatta una scommessa con se stessi e rispetto ai propri elettori, al proprio bacino di riferimento - chiamiamolo così l'unica umiltà che bisogna riconoscersi e che bisogna praticare è l'umiltà della responsabilità. Ci si può dimettere dalle funzioni, ma non dalla responsabilità che quella funzione reca. E se si fa il parlamentare, si è uno dei 1.000 italiani che sono parlamentari della Repubblica e si deve cercare di fare il meglio che si riesce a fare.

che la legittimazione di chi si oppone è identica alla legittimazione di chi invece lavora sul testo, cercando di fare il miglior lavoro possibile, nel rispetto delle regole e delle istituzioni e in adempimento del dovere cui ciascuno di noi è tenuto.

Poi, ovviamente, a qualcuno di voi probabilmente sembrerà poco significativa questa difesa del Parlamento,

sia rischioso, molto rischioso. Evidentemente abbiamo troppa fiducia nelle istituzioni e nella nostra democrazia, salda, fortunatamente, molto salda, per poter correre questo rischio. Come dicevo ai colleghi in premessa, ho tentato di raccogliere ancora gli echi del dibattito su alcuni aspetti e so che uno degli aspetti portato in discussione soprattutto dai colleghi che si oppongono a questo testo è quello della delimitazione dei poteri del Comitato e, in particolare, della necessità che il Parlamento conservi piena ogni sua attribuzione, ogni suo potere. raccogliendo queste ulteriori suggestioni, ho presentato alcuni emendamenti che ancora una volta precisano l'ambito, definito

Grazie, immagino verrà stabilito un termine per la presentazione di subemendamenti, in maniera da poterne affrontare la discussione e la votazione. Voglio davvero ringraziare tutti i colleghi per la collaborazione e ancora una volta lasciatemi ringraziare per l'eccellente collaborazione gli Uffici del Senato.

nel cuore del parlamentarismo e, in particolare, nel cuore del rapporto tra il potere esecutivo e il potere legislativo. Noi stiamo iniziando un procedimento di revisione costituzionale. Stiamo modificando la nostra Costituzione; la stiamo modificando

perché queste modifiche sono parte del programma di un Governo molto particolare che ci siamo dati in un momento di difficoltà istituzionale; di un Governo che ha deciso di investire la sua stessa esistenza su questa partita e addirittura di darsi un Ministro per le riforme costituzionali. Lo stiamo facendo sapendo che la caratteristica del regime parlamentare - del nostro regime parlamentare è quella per la quale i due poteri, quello esecutivo e quello legislativo, hanno uno spazio di autonomia e di separatezza ma anche un necessario collegamento che è garantito dal voto di fiducia e che rappresenta la caratteristica del regime parlamentare. È ciò che lo differenzia da una parte

nel momento in cui vi è una modifica della Costituzione da fare, soprattutto nelle contingenze storiche date. Dunque, io ho assunto questo periodo - quello trascorso dal momento della presentazione in quest'Aula del disegno di legge da parte del Governo ad oggi, quando si è conclusa la discussione generale come un tentativo di trovare la giusta calibratura tra autonomia e collegamento, tra separatezza e necessaria collaborazione.

Mi rivolgo al collega Crimi, del quale apprezzo sempre la chiarezza degli interventi. È vero: questa legge è una legge del Governo,

rispettando anche alcuni aspetti che magari si sarebbero potuti chiarire fin dall'inizio e che invece, giustamente

da un canto trent'anni di dibattito su questi temi, che ci hanno consentito di sviscerare qualsiasi aspetto dal punto di vista tecnico; dall'altro, il fatto che che ci si trova di fronte ad una crisi, quella che stiamo vivendo, che ormai sta durando più del tempo di una guerra mondiale del Novecento; che sta cambiando non soltanto la cultura politica, ma anche molte delle categorie culturali e politiche con le quali noi siamo abituati a convivere e che ci porta a dire che nulla

di un rapporto vissuto su barricate contrapposte o quantomeno distinte, sia che si aderisse alla cultura del libero mercato sia alle interpretazioni marxiste e persino a quelle corporative.

Significa proiettarci nel nostro compito di riforma in avanti, considerando le sconfitte e anche il lavoro che abbiamo alle spalle. dei 18 mesi sia stata un elemento di consapevolezza da parte del Parlamento. Perché la centralità parlamentare non può essere soltanto invocata nelle Aule: la centralità parlamentare si deve anche nutrire della consapevolezza di ciò che c'è nel Paese, di ciò che il Paese si aspetta. E su questo terreno si aspetta che non si perda tempo, che non ci sia un altro rimando. Credo che a tal riguardo tutte le forze politiche debbano fare una analisi autocritica sul modo con cui ci si è approcciati a questo tema nella scorsa legislatura. Probabilmente i risultati elettorali di qualche mese fa sono stati anche il frutto di una sordità che magari, a volte, si è avvantaggiata anche di una declaratoria di centralità del Parlamento che non abbiamo saputo tradurre nei fatti. Ma se quei 18 mesi sono stati un elemento di equilibrio e - se si vuole - di responsabilità, per contemperare il fatto che stiamo modificando la Carta costituzionale del nostro Paese, la Carta fondamentale, fondamentale, e il fatto di non poter dare nemmeno l'impressione di voler cincischiare con le riforme - come è stato scritto

il Governo ha assecondato il dibattito che si è svolto in Commissione ed è arrivato, insieme ai senatori della 1a Commissione, a definire una scadenza differente rispetto a quella

prevedere una ripartizione dei compiti. Se è del Parlamento utilizzare al meglio il tempo che gli si è interamente consacrato, è del Governo garantire che quel crono programma che ci si è dati in piena libertà venga rispettato e che le riforme non siano ancora una volta uno strumento per allungare i tempi, e non importa dei tempi della legislatura o di quelli della vita del Governo. Noi sappiamo, mai come in questo caso, che sia la legislatura che l'attuale Governo devono stare in piedi fino a che servono

dei Titoli I, II, III e V, era evidente che il Governo avrebbe potuto prevedere

Non certo, colleghi, perché non ci sia la consapevolezza, anche nel Governo, che il problema del rapporto tra il potere giudiziario e il potere politico sia uno dei capitoli più importanti più importanti di una riforma dello Stato. Si possono avere i giudizi più diversi, ma sul fatto che ci sia la necessità di intervenire su un aspetto che ha determinato la fine - e direi anche una fine traumatica - di Governi sia di centrodestra che di centro‑sinistra, credo che nessuno di noi abbia dubbi. Ma proprio perché vi è tale consapevolezza, nessuno può credere che questo tema lo si volesse trattare attraverso un emendamento presentato di soppiatto. Si tratta di un grande tema cui dovremo confrontarci e sul quale si aprirà il confronto all'interno del Governo. Abbiamo anche una traccia precisa di riforme possibili

tra esponenti provenienti dal centrodestra, dal centro e dal centrosinistra, ma persino con un rappresentante della scuola della magistratura. È quello il programma al quale guardiamo e nessuno ha mai inteso introdurre di soppiatto qualcosa di differente all'interno di questo procedimento, per il rispetto che si deve ad un procedimento di revisione costituzionale, ma anche - consentitemelo - per il rispetto che si deve alla rilevanza del tema del tema dei rapporti tra potere giudiziario e potere politico. Non è argomento che si può trattare attraverso un emendamento. Anche in questo caso, al netto di qualche polemica giornalistica che è il tentativo a volte di agitare l'acqua all'interno di un bicchiere, si è arrivati non solo a capirsi ma anche a trovare la definizione migliore. Così come, per quanto riguarda la legge elettorale,

che non ha un rapporto di obbligatorietà con la forma di governo e con l'impianto complessivo del sistema politico, ma ha

del parlamentarismo, quel Walter Bagehot che considerava il sistema elettorale come uno degli elementi fondamentali del sistema di Gabinetto.

che abbiamo compiuto tutti insieme, è l'aver voluto caricare sulle spalle troppo gracili della legge elettorale il peso di un'intera riforma del sistema. Si tratta di un vizio antico, che è della storia d'Italia e che affonda le sue radici addirittura nella stagione dell'Italia liberale, quando gli oppositori di Giolitti avrebbero voluto farlo fuori cambiando la legge elettorale e, poi, addebitato ingiustamente alla proporzionale il danno di aver portato un regime autoritario. Questo vizio antico, in tempi più recenti è diventato addirittura parodia. Basti pensare che soltanto qualche decennio fa, c'è chi diceva che il toccasana per il nostro sistema sarebbe consistito nella eliminazione delle preferenze. Si è tenuto anche un *referendum* su questo. persone, qualche decennio più tardi, in alcuni casi, ritengono che il toccasana possa essere la reintroduzione delle preferenze. Diciamo che la legge elettorale è un pezzo importante di un più complessivo

importante si sia raggiunto in Commissione, non soltanto nel clima, ma anche nel dialogo che si è svolto con le opposizioni. Non ho ancora sentito - per onestà mi piacerebbe che qualcuno dicesse una parola - una considerazione sul fatto che, quando questo dibattito è iniziato, si parlava di una convenzione in cui fossero presenti parlamentari e cosiddetti laici, i quali hanno una fonte di legittimità - in questo caso, sì, si deve scomodare la categoria della legittimità - molto differente. Infatti, i parlamentari sono legittimati dal voto popolare, mentre gli altri sarebbero stati nominati. Questa convenzione avrebbe dovuto avere poteri redigenti

giorni un po' di acqua sotto i ponti sia passata, e forse, se qualcuno ha veramente a cuore la centralità del Parlamento, lo dovrebbe riconoscere e dovrebbe riconoscere anche anche che il Governo ha fatto qualcosa perché questa centralità si affermasse. Oggi siamo in presenza di qualcosa di molto diverso, che chiamerei un «138 rafforzato», perché le norme sul *referendum* e sul fatto che il *referendum* possa riguardare materie omogenee e autosufficienti sono una garanzia in più e non una garanzia in meno: forse questo dovrebbe essere riconosciuto. Però, al di là di questo riconoscimento che è mancato - ma c'è sempre tempo e finché c'è tempo c'è speranza -, vorrei evidenziare anche come, sulla necessità di integrare il dibattito parlamentare con l'utilizzo anche di nuovi mezzi di comunicazione di massa, si è fortemente discusso e - credo - si siano fatti passi avanti notevoli. Mi fa piacere il riconoscimento che è venuto dal senatore Crimi all'iniziativa del Governo. Se il Governo si è fatto carico di quella iniziativa, così come si è fatto carico di consultare 35 docenti docenti di materie inerenti a questo tema in un tempo nel quale il Parlamento non lavora nel merito delle riforme, lo ha fatto anche per rispettare la centralità del Parlamento. elementi, infatti, sono un modo per portare il dibattito fuori dal Palazzo, per cercare di arricchirlo e di offrirlo alla riflessione del Parlamento, che però deve essere libero di farne quello che vuole, di prendere in considerazione i diversi aspetti, di considerarli parzialmente o anche di metterli da parte, sia che essi arrivino dalla sapienza di alcuni professori universitari sia che arrivino dalla rete, perché la centralità del Parlamento o vale sempre o non vale mai. Noi crediamo debba essere rispettato il fatto che la Commissione possa lavorare senza interferenze esterne. È a questo proposito che abbiamo contribuito ad un ordine del giorno che intende quegli strumenti come un arricchimento del parlamentarismo, perché il parlamentarismo nella sua nella sua storia si è spesso modificato. Non era lo stesso quando i Parlamenti nacquero e quando i partiti erano poco più che *club* elitari; diventò una cosa differente quando le masse entrarono nella vita pubblica e i partiti diventarono partiti di integrazione di massa; e si modificò ancora quando nacque la stampa nazionale, poi la radio e la televisione. Ora siamo ad un altro tornante, che è giusto considerare perché la forza del parlamentarismo è proprio quella di sapersi adeguare, di essere il sistema più elastico che è stato fin qui ideato nella storia della politica. Ma il parlamentarismo ha alcuni principi

all'ascolto, uscire dal palazzo e dalla retorica del palazzo, ma allo stesso tempo dobbiamo rispettare quei princìpi del parlamentarismo che valevano ieri e valgono oggi. Perché le condizioni quali quei princìpi si adattano cambiano, ma i principi di fondo no. Il senatore Compagna ha detto, con un'immagine che Parlamento è una bicicletta e il Ministero dell'economia è un carro armato. Io non so se la metafora sia perfetta, ma, se posso riprenderla,

abbiamo superato un momento difficile e abbiamo compreso non soltanto le proporzioni ma anche la calibratura dei rispettivi interventi e dei rispettivi spazi di autonomia. Per questo, colleghi, chiudo il dibattito con molta più serenità di quella che avevo il giorno in cui ho presentato in quest'Aula il disegno di legge costituzionale. Se non è un buon inizio, quantomeno è un buon auspicio. *(Applausi

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In ordine agli emendamenti il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.42, 2.36,

4.300, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta». Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli ordini del giorno G105, G107, G108, G113 e l'emendamento 2.100, in quanto anticipano questioni di merito attinenti a specifiche riforme, risultando pertanto estranei al contenuto del disegno di legge costituzionale in esame, che reca disposizioni per l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali, introducendo norme di carattere procedurale. La Presidenza dichiara altresì inammissibile l'emendamento 9.100,

Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Allo scopo di garantire una discussione e una trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno unitaria, le chiediamo, apprezzate le circostanze, di rinviare alla seduta di domani mattina il voto.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi che state lasciando l'Aula (e me ne dispiaccio), è incredibile come in questo Paese ci si abitui a tutto. I disastri sono così tanti e di tale entità che un terremoto di 5.2 gradi della scala Richter quasi non fa notizia. Noi del Movimento 5 Stelle, comunque, non ci vogliamo abituare al degrado e al disagio, e segnaliamo e denunciamo sempre. Ebbene, nella mia zona di provenienza, l'alta Toscana, il territorio negli ultimi tempi è stato oggetto di diverse catastrofi, fino ad arrivare

Toscana, il territorio negli ultimi tempi è stato oggetto di diverse catastrofi, fino ad arrivare al terremoto del 21 giugno, che ha registrato il livello altissimo di magnitudo 5.2. Anche questa notte c'è stata un'ulteriore scossa del 3.5, e un'altra poche ore fa. I paesi della Garfagnana e della Lunigiana sono in ginocchio. Il sisma che ha iniziato a terrorizzare la cittadinanza dal primo giorno ad oggi ha fatto riscontrare più di 1.600 scosse, ed alcune fortissime (da 4.2 e 4.4), come quella che due domeniche fa ho avuto modo di avvertire proprio mentre stavo visitando la zona. Il paese di Regnano e tutti i dintorni hanno tremato all'inverosimile, praticamente il cuore dell'epicentro. Secondi interminabili, che vi assicuro non si dimenticano. Avete presente un urlo che viene dal centro della terra? Alla fine non si capisce se terrorizzano di più le cose che si muovono intorno e crollano o il grido della terra che strazia i timpani. E quando tutto intorno si alza la polvere, allora comprendi meglio il perché degli sguardi impauriti dei cittadini. Nei Comuni di Fivizzano, Casola, Minucciano e Giuncugnano le persone vivono ogni attimo come il momento in cui può verificarsi una nuova scossa. A Monzone, Gragnola, Codiponte, Equi Terme, Vigneta e Regnano gli abitanti, ormai rassegnati, dormono nei centri allestiti dai volontari per le emergenze o nelle loro auto. La maggior parte della popolazione è costituita da persone anziane, soprattutto donne, che hanno abitudini ben radicate e un attaccamento al territorio comprensibile; infatti molti di loro hanno animali da accudire e campi da coltivare. Pertanto è scontata la loro diffidenza a trasferirsi in centri RSA. La Lunigiana e la Garfagnana sono località incastonate all'interno dell'Alta Toscana, territorio legato da una forte tradizione rurale, paesini che sembrano presepi, con tanto di borghi, castelli e pievi romaniche di rara bellezza. Dalle prime dichiarazioni del capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che aveva inizialmente utilizzato la parola "non evento" per catalogare tali avvenimenti, si pensava che il sisma non avesse avuto gravi conseguenze. Ebbene, oggi, dopo aver doverosamente visitato, certo non esclusivamente dall'alto di un elicottero, questi Comuni e le loro singole frazioni, è evidente il disastro abitativo; infatti alcuni borghi sono dichiarati zona rossa. Tra Lunigiana e Garfagnana ad oggi sono inagibili quasi 1.000 abitazioni. Ieri il senatore Barani diceva di rimpiangere Guido Bertolaso. Noi oggi diciamo che la Lunigiana, ha già abbastanza disastri così di suo *(Applausi dal Gruppo di non veder mai più persone inadeguate in azione, né promesse *spot* di dentiere nuove alle vecchiette da parte di politici patetici. Per tale disastro è stato decretato pochi giorni fa lo stato di emergenza: arriveranno i 5 milioni di euro promessi dal Governo? E, se sì, quando? Abbiamo comunque un dubbio: queste risorse non saranno sufficienti a soddisfare gli impegni per la ricostruzione, visto che il sisma sta continuando in maniera incisiva e in maniera incisiva e i danni stanno aumentando di giorno in giorno. I cittadini colpiti dal sisma vorrebbero tornare alla normalità. Solo se verranno adottate realmente tutte le misure necessarie, si potrà dire di aver fatto il nostro dovere; quindi ricostruzione subito e messa in sicurezza degli edifici. Il Movimento 5 Stelle vigilerà e non lascerà soli gli abitanti, così provati, di Lunigiana e Garfagnana. Grazie, signor Presidente.